Grazie

Grazie L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B

Poiché la Commissione bilancio non ha ancora dato il parere sull'emendamento del Governo 1.1000 e si è convocata per esprimere tale parere alle ore 10,

una nuova finestra"). A nome dell'Assemblea saluto la famiglia del defunto ispettore capo della Polizia di Stato Filippo Raciti, che ci fa l'onore di essere in tribuna*.

la parte fondamentale dell'emendamento 1.1000 del Governo; ciò, appunto, in ragione dell'*iter* che ha visto l'approvazione in Commissione degli emendamenti senza il preventivo vaglio della Commissione bilancio e poi la proposizione in Aula dell'emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia. Pertanto, ci siamo limitati ad una valutazione dell'emendamento 1.1000, presentato nei tempi consentiti dalle circostanze di fatto. La maggioranza della Commissione ha ritenuto sostanzialmente osservate le norme di copertura dell'emendamento in questione. In realtà, a seguito dell'esame che le norme appaiono coperte in alcuni casi con riduzioni di autorizzazioni di spesa, in altri con tagli delle tabelle entro limiti che la Commissione bilancio di solito ritiene totalmente accettabili. Ciò consente alla maggioranza della Commissione di esprimere un parere favorevole sotto i profili di copertura all'emendamento in questione. Notiamo con particolare soddisfazione che - lo ribadisco - l'emendamento è il frutto dell'*iter* parlamentare che fin qui si è svolto del testo presentato dal Governo e del lavoro della 1a Commissione, senza l'inserimento di nuove materie, che avrebbero comportato una nuova relazione tecnica da parte del Governo. Ciò non si è reso necessario per le ragioni che ho poc'anzi espresso. I colleghi dell'opposizione hanno concentrato le loro osservazioni critiche sostanzialmente su tre aspetti. Il primo aspetto è di carattere generale ed è quello della ristrettezza dei tempi, che non ha consentito ai colleghi dell'opposizione un esame partito di tutti gli emendamenti e, di conseguenza, dei profili di copertura finanziaria di ciascuno di essi. I tempi sono stati ritenuti dall'opposizione (non senza qualche ragione) molto ristretti per la disamina specifica del testo.

è un'espressa previsione di invarianza degli oneri per una parte di quell'articolo,

presentata, e un piano specifico, perché a loro avviso si tratta di una norma che presenta profili di onerosità non adeguatamente coperti.

prima avevo avuto solo delle anticipazioni da parte di qualche fortunato che ieri sera era riuscito ad averne una copia. Ora, escludendo che i senatori debbano svolgere il loro lavoro senza supporti telematici dalle 10 di sera alle 6 di mattina,

compreso il relatore, forse uno dei pochi privilegiati che sa esattamente cosa c'è scritto in questo maxiemendamento, a dire che andremo a votare,

nemmeno le mille proroghe come da titolo, ma da sempre viene usato come strumento e veicolo di normative le più diverse.

non voglio riprendere i temi della polemica degli scorsi due giorni, se non per evidenziare che si è aperto un dibattito nel Paese, a partire da un episodio che mai avrebbe dovuto prestarsi ad essere usato per tale fine, su chi comanda, chi ha i poteri, chi riesce a decidere, eccetera. Per

ma anche di esame approfondito di certi emendamenti pur di rispettare i tempi dell'Aula e - voglio essere chiara, signora Presidente - non dare neanche una possibilità di alibi al Governo per chiedere la fiducia. Nonostante questo,

di una sospensione non di ore, ma di trenta minuti. Se poi anche questo spazio di riflessione e di approfondimento deve essere impedito, francamente resto basito, signora

conferma altresì che c'era un accordo per cominciare le dichiarazioni di voto alle 12,30. La Presidenza è consapevole della ristrettezza dei tempi.

richiamava anche il senatore Belisario, anch'io faccio un'osservazione di grande metodo politico‑istituzionale. Noi svolgiamo un dibattito su un così chiamato maxiemendamento, che effettivamente è giunto

lettura e interpretazione laddove il testo di riferimento avesse avuto un filo conduttore piuttosto definito. Questo provvedimento, chiamato per comodità milleproroghe, è francamente

hanno contraddizioni e richiami spesso illeggibili. Svolgo questo intervento condizionato dalla mannaia del voto di fiducia, perché

305 milioni di euro sono appannaggio di quelli che definiamo contributi indiretti, cioè le tariffe postali agevolate, che per lo più vanno ai grandi gruppi editoriali quotati in Borsa:

per tanti giornali, ivi compresi quelli di partito, che insieme a tanti altri fogli, che qui non sto a citare perché c'è già stata occasione di farlo, compongono un mosaico di circa un centinaio di soggetti editoriali che corrono seriamente il rischio, non ipotetico ma purtroppo molto reale, di vedersi tagliare la propria futura esistenza.

che qualcosa sia cambiato, ma non la certezza, perché l'effettiva congruenza di quel fondo va chiarita in modo esplicito e non informale in questa stessa Aula, augurabilmente in sede di riepilogo del dibattito

per sua natura temporaneo ai fini di aggiustamento e correzione della legislazione in vigore, mediante varie forme di modulazione di termini e di scadenze. Il Governo, oltre ad operare in misura sempre più rilevante, se non esclusiva, attraverso la decretazione di urgenza, aggiunge in questo decreto l'operazione di prorogare termini, con un effetto improprio di sistemazione della legislazione vigente. Tutto ciò con l'aggravante della fiducia, pur essendoci tutto il tempo per discuterne. Ci troviamo infatti di fronte ad una sorta di ordinaria attività di normazione svolta dal Governo amministrazione. La stessa amministrazione che, non rispettando i termini per gli adempimenti, nell'immediatezza dello scadere ne dispone la proroga con proprio decreto, accrescendo così l'incertezza degli operatori dei diversi settori e dei destinatari delle norme in generale circa l'effettiva necessità di conformarsi ai termini scritti nelle leggi, in vista di continui e sistematici rinvii. Per quanto riguarda il settore lavoro, siamo soddisfatti che nel maxiemendamento non siano stati inseriti i due emendamenti della Lega approvati in Commissione affari costituzionali. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti 32.5 e 32.6 che, modificando il testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (approvato dal Governo Prodi lo scorso aprile), andavano pesantemente ad incidere sulle necessarie misure poste in essere nella scorsa legislatura a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Purtroppo, invece, dobbiamo constatare la conferma dell'emendamento del Governo con il quale si provvede a prorogare di un altro anno (dal 2009 al 2010) il termine per l'emanazione dei decreti che il Governo avrebbe dovuto adottare per disciplinare la normativa sulla sicurezza in relazione a determinati comparti. Mi riferisco alle Forze armate e di polizia, al Dipartimento dei vigili del fuoco, al soccorso pubblico e alla difesa civile, ai servizi di protezione civile, nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, a quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, alle università, agli istituti di istruzione universitaria, agli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, alle organizzazioni di volontariato e ai mezzi di trasporto aereo e marittimo. Inoltre, il Governo proroga ancora di un anno il termine per l'adozione dei decreti necessari a consentire il coordinamento della disciplina recata dal testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con la normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale, per il settore delle navi da pesca e per l'armonizzazione delle disposizioni tecniche in tema di trasporto ferroviario. In questi giorni ci avete accusato di essere cultori della morte. Ma che cultori della vita siete voi, che non siete minimamente interessati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, malgrado le migliaia di morti bianche e gli innumerevoli incidenti che avvengono ogni anno? Con il milleproroghe volete posticipare di un anno i tempi per adeguarsi alle nuove norme sulla sicurezza; tutto rinviato di un anno, in barba a quello che purtroppo accade ogni giorno in Italia, dove ogni sette ore c'è una vittima del lavoro. Cadono così nel vuoto gli appelli del Presidente della Repubblica e della CEI, che chiedono luoghi di lavoro a misura d'uomo:

Signora Presidente, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, avrei preferito intervenire nell'ambito della discussione sui singoli articoli, per presentare alcuni emendamenti migliorativi del nostro Gruppo. Invece, ancora una volta dobbiamo accontentarci di essere spettatori passivi delle decisioni del Governo. Ogni volta ‑ e ce ne sono state davvero tante che ci viene chiesta la fiducia stigmatizziamo la pericolosità e l'incongruità di questo modo di operare. Diventa fin troppo facile ripetere all'infinito che con la richiesta di fiducia si esautora il ruolo del Parlamento, che viene meno il confronto nel merito delle questioni tra maggioranza, opposizione e Governo. Sono critiche destinate a rimanere senza risposta; anzi si fa ricorso alla fiducia anche per un provvedimento che non tratta di questioni rilevanti dal punto di vista politico, ma che attiene alla quotidianità delle cose ed è proprio per questo che ci si attendeva un'apertura da parte del Governo ad accogliere anche in questa sede alcuni emendamenti migliorativi. Già in Commissione si è proceduto ad approvare alcune modifiche da noi proposte, che avevano come unico obiettivo quello di dare risposta alle aspettative dei cittadini. Purtroppo adesso ci è preclusa tale possibilità, la possibilità di incidere ulteriormente, e non si tratta di pregiudizi, di posizioni preconcette: si tratta esclusivamente di buonsenso,

il testo contiene dispositivi anche utili, ma tanti interventi che non possono essere assolutamente condivisi. Non entrerò nel merito dei singoli articoli, mi soffermerò solamente su alcuni aspetti che destano preoccupazione. Uno dei più contrastati è sicuramente il tema della sicurezza sul posto di lavoro. Nelle ultime settimane mi sono occupata specificatamente di questo tema, dopo due incidenti mortali in una sola settimana nella mia città, Trieste. Come possiamo leggere ogni giorno, si tratta di un fenomeno che sta crescendo, è un fenomeno che con l'acuirsi della crisi potrebbe assumere aspetti ancora più preoccupanti per ciò richiederebbe un'attenzione particolare del Governo. Invece il decreto prevede la proroga dei termini per l'assolvimento di alcuni obblighi da parte dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Per fortuna, come abbiamo visto, è stato è stato depennato l'emendamento approvato in Commissione su questo tema. In questo modo, invece di alzare il livello di guardia sull'argomento si va nella direzione opposta. Che dire poi di talune proroghe, come ad esempio quella relativa alla *class action*? Ci si aspetterebbe, in questo momento di grave crisi economica che colpisce in particolare le famiglie di consumatori, l'attuazione di tutte le misure di tutela

sulle stabilizzazioni degli enti di ricerca: si tratta di temi di grande portata ed attualità, che andrebbero discussi a parte, con norme specifiche e non con interventi di parte ed *una tantum*. *una tantum*. Devo dire, invece, di avere appreso con soddisfazione che talune nostre proposte fatte in occasione della finanziaria sono state recepite in questo milleproroghe; in particolare, vorrei sottolineare il fatto che sono stati i fondi per la minoranza slovena tagliati dalla finanziaria: mi riferisco al comma 11 dell'articolo 41 che prevede il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di questi fondi. Vorrei infine ribadire che esprimeremo voto contrario sulla fiducia ed ancora una volta rimarcare che purtroppo queste discussioni avvengono in un'Aula che è praticamente deserta, soprattutto da parte della maggioranza.

Ciò detto, ci sono altre cose che in questo maxiemendamento mi preoccupano. È rimasto infatti l'articolo 10, che rimanda le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero,

Non rispettare le scadenze naturali di organismi di rappresentanza non è mai un buon segnale. Se poi questo segnale lo avviciniamo a quel che registriamo in questo Parlamento, questo Parlamento, che sembra venga vissuto come un fastidio del sistema e del funzionamento del nostro Stato, Stato, allora dovremmo riflettere. Ma più che riflettere noi dell'opposizione, perché i numeri sono quelli che sono, dovrebbero riflettere i colleghi della maggioranza. anche il modo di operare. Basta vedere ieri sera le ore che abbiamo passato seduti ad aspettare: sospensione, non sospensione... Non è un bel vedere. Non è un gran bel segnale di rispetto, da parte del Governo, del Parlamento, un pezzo

In ultimo, volevo ricordare al Governo un aspetto. Il decreto milleproroghe, mi è stato spiegato nei pochi anni che ho passato in questo Senato, serve a correggere i naturali errori che si commettono in un anno. il 2009, per ciò che riguarda gli italiani all'estero, non ha deciso solo tagli drammatici che ci portano alla chiusura di tutti i corsi di lingua e cultura italiana nel mondo

aver lasciato l'ICI sulle case degli italiani all'estero e che l'avrebbero corretto. Allora vorrei ricordare alla memoria del Governo che gli unici cittadini italiani che pagano l'ICI non sono i milionari che noi, con il nostro Governo, avevamo escluso ma gli operai italiani che si sono fatti una casetta per tornarci in vacanza. Non solo ci vivono tre settimane o un mese l'anno, ma sono rimasti gli unici a pagare l'ICI.

e non vivono molto bene questo momento della politica italiana. Ma i vostri elettori veramente non sanno più dove sbattere la testa. Cercate di ricordarvi qualcosa ogni tanto.

il ricorso al voto di fiducia sta diventando una prassi inaccettabile. Il Governo, forte di una maggioranza schiacciante, continua a ricorrere al voto di fiducia ritenendo inutile orpello le Assemblee e le prerogative dei parlamentari. Noi non possiamo neppure entrare nel merito, lo ha detto anche il nostro Capogruppo, Belisario, non possiamo esaminare quel che è

Si ritiene che il Parlamento sia un intralcio al decisionismo e all'azione di Governo. Voglio solo ricordare che, probabilmente perché non vi fidate della maggioranza, questo combinato disposto, oltre a comprimere i tempi, costituisce un *vulnus* perfino all'articolo 81 della Costituzione, per quanto attiene alle coperture finanziarie. Ma sul punto mi soffermerò Cosa contiene questo maxiemendamento che in poche ore dobbiamo esaminare e poi votare? Di tutto e di più. Dal trattamento accessorio del personale della pubblica amministrazione, alla promozione di funzionari del Ministero degli affari esteri, a norme destinati agli agricoltori sardi

la norma a favore dei tassisti per la disciplina del servizio di autonoleggio, il finanziamento per la prosecuzione dell'autostrada ferrovie alpine, gli arbitrati (ancora una volta volta il divieto di arbitrato viene prorogato) e una serie di altre misure. Nel breve tempo che ho a disposizione mi soffermerò sull'azione di classe, una norma conquistata in quest'Aula un paio di anni fa con un solo voto di scarto perché richiesta dai cittadini, dai consumatori, dai risparmiatori frodati dalle banche, tartassati dalle compagnie di assicurazione, norma che doveva entrare in vigore il primo luglio del 2008, mentre è stata rinviata

dei consumatori. Considero quindi gravissimo il rinvio alle calende greche dell'azione di classe, lo considero un *vulnus* ai diritti dei cittadini e dei consumatori; lo ripeto, un milione di risparmiatori frodati che non possono avere accesso alla giustizia a causa dei lunghi tempi della giustizia, mentre

al *business plan*) sul totale dell'operazione. Siamo indietro del 20 per cento. L'*investor report* riporta le risposte degli enti sollecitati a vendere: «problemi di contenziosi» (ENPALS, che nel trimestre ha mancato gli obiettivi del 100

avrebbe potuto rappresentare lo strumento per apprestare una serie di risposte ai problemi, ormai troppi, dei comparti dell'agricoltura e della pesca che attendono una soluzione ed è soprattutto su tali tematiche che intendo invece no! Salvo un paio di eccezioni, di cui correttamente riferirò, anche questa occasione è stata mancata dal Governo. Anche questa, dico, perché ve ne sono state altre, importanti e certamente più specifiche che avrebbero costituito - per definizione - la concreta opportunità per prendere atto della condizione di sofferenza del settore primario, ormai in crisi strutturale, come il Partito Democratico aveva da tempo evidenziato:

il maxiemendamento al decreto proroga termini sul quale il Governo, con procedura ormai abituale, che comprime, fino a mortificarlo, il ruolo del Parlamento, pone la questione di fiducia, con riguardo alle problematiche del comparto primario prevede semplicemente, come da più parti era stato sollecitato (per quanto ci riguarda, emendamenti della senatrice Bertuzzi e del senatore Legnini), l'esenzione dall'ICI sulle unità immobiliari aventi requisiti di ruralità e pertanto non non considerati fabbricati. Di ciò naturalmente prendiamo atto con piacere proprio perché la questione era sta più volte anche da noi del PD sollevata. All'articolo 3 viene introdotta una disposizione secondo la quale si prevede il controllo parlamentare sulle nomine presso gli enti vigilati dal Ministero per le politiche agricole. È una apprezzabile misura di trasparenza; occorrerebbe tuttavia chiarire le modalità di queste nomine. Chiediamo quindi che su tutto ciò ci sia un ulteriore ed urgente approfondimento, in omaggio al principio di evidenza pubblica, che dovremo aver aver cura di far osservare, e di accorta selezione per merito della competenza specifica. Il maxiemendamento esclude invece, contrariamente a quanto il Partito Democratico aveva proposto con propri emendamenti, il beneficio del canone ricognitorio a favore della pesca e dell'acquacoltura, l'interpretazione autentica del contenzioso INPS relativamente ai contributi SCAU, la proroga dal 31 marzo al 31 dicembre 2009 delle agevolazioni previdenziali nelle aree svantaggiate e nelle zone montane. Il Governo aveva poi presentato alla Camera un emendamento contenente disposizioni in materia di ricostruzione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna. lettura del senatore Lanutti: anch'io, come lui, ho avuto tra le mani ieri sera dopo le 21 il testo del maxiemendamento e a me non pare di avere scorto questo provvedimento. Era una questione delicata e aperta, che si trascina dai primi anni '90 e che avrebbe trovato soluzione - ahimè -soltanto in prossimità delle elezioni regionali. Come Partito Democratico avevamo semplicemente rilevato che sarebbe stato ingiusto non prevedere analoghe agevolazioni per le imprese agricole operanti nel resto del territorio nazionale.

Da quanto esposto fin qui si evince nitidamente come, al di là di qualche rara eccezione, permanga da parte del Governo una sostanziale e reiterata disattenzione verso i problemi della agricoltura e della pesca, la stessa disattenzione che cogliamo nel vedere di fronte a noi i banchi vuoti della maggioranza. Cogliamo la presenza soltanto di pochi colleghi, che evidentemente avvertono il senso della loro responsabilità

di cui è prima firmataria la collega senatrice Pignedoli, sullo stato di crisi del settore agroalimentare e della pesca, che prelude ad un disegno di legge su analogo tema. Rassegnerò l'intervento agli atti, signora Presidente, perché vi erano alcune specificazioni che ho omesso per rispettare i tempi. *(Applausi

come hanno sottolineato i colleghi intervenuti prima di me, abbiamo avuto tempi strettissimi per esaminare il maxiemendamento

ai lavoratori in pensione sono da tempo arrivate lettere ed in alcuni casi è stata sospesa l'erogazione della pensione. Stiamo parlando di persone che vivono di pensione.

i cosiddetti ex co.co.co, che si trovano disoccupati a partire dal dicembre 2008. A Genova ci sono 200 lavoratori dell'università, di professionalità di rilievo - bibliotecari, informatici,

Consorzio autonomo del porto e l'INPS stessa, con tanto di protocolli sottoscritti e controfirmati. Vi rappresento quindi la situazione di una città che, da questo punto di vista, sia per il problema di pensionati che vivono con un unico reddito,

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, per quanto mi riguarda si tratta di una fiducia tecnica al Governo che si colora, nella circostanza, di accentuati contenuti politici. La definisco così perché, sul piano tecnico, non c'è dubbio che il maxiemendamento si presenta come apprezzabile e corretto: soccorre ad esigenze reali, è innegabile. L'opposizione può anche stiracchiare qualche tesi facendo il suo mestiere, ma sono tutte norme sostanzialmente giuste che vengono incontro ad esigenze reali di importanti settori del Paese. a titolo di esemplificazione di quel che dico, parlare dell'articolo 2, relativo alla non applicazione agli enti locali, a certe condizioni, di conseguenze relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, tema di grandissimo rilievo per gli enti locali governati da sindaci di qualsiasi versante politico. Potrei anche parlarvi dell'articolo 7-*bis*, dove si stabilisce che con il concorso delle organizzazioni sindacali è possibile prospettare criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa. È un tema di straordinario ed eccezionale rilievo, ne abbiamo parlato tante volte in entrambi i versanti politici. Potrei parlarvi dell'articolo 21, volto a continuare a garantire l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza

di persone che si venivano a trovare in queste delicate situazioni, anche con conseguenze fiscali di grande rilievo. Potrei parlarvi dell'articolo 35, che attiene al personale degli enti di ricerca, con problemi che abbiamo affrontato tante volte in termini assai allarmati

al fondo per interventi strutturali di politica economica, con tante conseguenze di carattere fiscale, che soccorrono anche alle scadenze per i contribuenti ed i loro consulenti, i quali ci hanno più volte richiesto questo tipo di interventi. Potrei parlarvi dell'articolo 44-*ter*, che reca disposizioni in materia di infrastrutture carcerarie, in cui con grande attenzione e sensibilità si interviene, così come con

nel provvedimento. Ognuno di noi, non lo neghiamo, si è infatti attivato per inserire delle norme che soccorressero a particolari, ma non particolaristiche, esigenze, che pur hanno un loro rilievo. Io stesso, che pur sono parlamentare della maggioranza governativa, sono stato firmatario di non meno di una quindicina di emendamenti (che non ho buttato là per caso),

fiducia tecnica, perché si tratta di rispettare dei tempi e delle cadenze rispetto ai quali questa enorme quantità di proposte di emendamento, provenienti da tutti i settori del Parlamento, avrebbe indubbiamente fatto fatto impelagare ciascuno di noi e l'Esecutivo in una controversa serie di esami e di problemi, da cui, anche come tempi, non si sarebbe usciti. Quindi, una fiducia tecnica motivata anche politicamente. Qui, onorevoli colleghi, non possiamo attardarci in disquisizioni tecniche, come se vivessimo fuori del mondo politico, senza tener presente che la seduta odierna segue ad altre sedute, partecipate con un calore ed una veemenza ben diversa da quella che ci può motivare ad un confronto tecnico su tali norme. almeno per quanto mi riguarda si tratta di un fiducia tecnica che coloro molto in termini politici. Sì, qualcuno di voi può anche ritenere che si sia fuori tema. Questo poco mi fa crucciare. quello che è accaduto nelle giornate trascorse è qualcosa che, al di là della procedura, dà alla maggioranza di Governo Governo l'autocoscienza delle grandissime responsabilità civili che su di essa gravano e che - la vogliamo dir tutta in questi tempi di ipocrisia buonista, che è il contrario del colloquio costruttivo motiva anche ad essere voi, colleghi dell'opposizione, e noi della maggioranza, ciò che siamo e che dobbiamo, anche in maniera contrapposta, essere, spiegandoci e presentandoci come tali all'opinione pubblica. Non c'è spazio per disorientamenti. Anche i migliori colloqui si radicano sulla corretta definizione delle rispettive identità e responsabilità. Questo è il mio modestissimo pensiero. Mi ha divertito un po' nei giorni scorsi vedere alcuni quotidiani che rappresentavano il modestissimo sottoscritto - troppo onore - e qualche altro collega quasi come gli avanguardisti di un assalto non certo fisico, ma perlomeno dialettico o veemente, nei confronti dell'opposizione del nostro emiciclo. La cosa mi ha molto divertito perché, sapete bene, di solito me ne sto al mio e mi diletto poco di confronti fisici; non mi esaltano e forse non ne ho neanche i numeri. Però non mi è dispiaciuto da quel punto di vista, perché si riferiva ad un confronto forte, anche un po' acerbo, che si era determinato a seguito dell'intervento

chi, invece, si sente ancora, tutto sommato, un galantuomo ed è qui per sostenere dei convincimenti. Onorevoli senatori, è arrivato il momento di vivere anche il clima giusto, la contrapposizione giusta, l'alternativa civile e corretta, perché la gente capisca chi fa le cose, per quale ragione e con quali ritorni utili o negativi. Ecco perché, con un clima di rinnovata chiarezza, bisogna affrontare, con consapevolezza politica, un voto di fiducia, che è cosa alta e importante, anche se si ripete per 10, 15, 20 volte. Non mi diletto della polemicuzza del dire sì; noi l'abbiamo posta 12 volte, ma voi l'avevate posta 24. Non m'interessa più di tanto dire se è stata tirata la corda nel porre la fiducia, scavalcando il Parlamento. Questo è un tema delicatissimo, ma non scomodiamolo in questa circostanza, sul milleproroghe, che è un difettuccio di tutti i Governi da 25 o 30 anni a questa parte. Scomodiamola per altri provvedimenti, per altri temi. della sovranità del Parlamento e del corretto equilibro, tutto in evoluzione, tra l'esecutivo e il legislativo. In questo caso, scomoderemmo importanti sistemi per un'occasione che, forse, vale meno la pena di altre circostanze. Ricordiamoci del clima,

di dilazione, *strictu sensu*, della vigenza di certe norme, altri, invece, sotto l'aspetto della proroga dei termini, tendono anche ad introdurre una qualche forma di normazione che non è strettamente riferita ai termini, se proprio vogliamo fare dell'esegesi pignola e critica. possiamo dire che si tratta di norme che ci mettono certamente nella condizione di affrontare vari nodi di carattere politico, sociale ed economico, con maggiore tranquillità, senza l'incombere di scadenze che avrebbero, di per sé stesse, un effetto negativo. Ecco perché ho motivato questa fiducia che sicuramente esprimerò a favore del Governo in termini tecnici, politicamente colorati e riempiti di significato politico. *(Applausi dal Gruppo

Signora Presidente, colleghi, il mio intervento sarà breve. In apertura, vorrei invitare i colleghi Lannutti e Micheloni - non ho il piacere di ricordare se nella scorsa legislatura erano in Aula con noi - ad andare a verificare quante fiducie aveva messo il Governo Prodi in dieci mesi e quante ne ha messe il Governo Berlusconi: credo che davvero il primo vincerebbe ampiamente questa classifica. Ma io intervengo solo ed esclusivamente per ricollegarmi all'intervento della collega Pinotti e sottolineare l'importanza e la gravità sociale della vicenda dell'amianto.

sociale. Non è giusto che costoro paghino, in una vicenda, come quella dell'amianto, che è costata tanto allo Stato italiano, ha visto anche un intervento del Governo Berlusconi nella legge finanziaria del 2003 e comunque allora aveva certi contorni che oggi non possono essere messi in discussione. All'INAIL è arrivata la richiesta di rivedere migliaia e migliaia di pensioni: non credo che pensionati che hanno da 65 a 70 o 75 anni, le cui aziende e i cui posti di lavoro non ci sono più, possano vedere messa a rischio la loro pensione e soprattutto vedersi anche richiesti

di inserirlo nel primo provvedimento utile che verrà calendarizzato, che a quanto pare, secondo quanto ricordava anche la collega Pinotti, è quello relativo agli incentivi per le case automobilistiche.

intervengo in relazione ad una modifica che riguarda contemporaneamente sia il settore giustizia sia il comparto sicurezza e che è per certi versi strabiliante, anche se ormai non ci meravigliamo più di nulla,

non soltanto a modificarla, ma a rettificare quanto la stessa Commissione giustizia e la maggioranza all'interno di essa avevano detto e votato a favore del Fondo unico giustizia. All'interno della Commissione, c'erano state una diatriba ed una grossa discussione, con tutta una serie di emendamenti, relativi alla destinazione del Fondo unico giustizia. Con particolare riferimento, si chiedeva, da parte nostra, come Partito Democratico, di destinare i fondi indicati appunto come Fondo unico giustizia soprattutto al settore giustizia e, in subordine, eventualmente al comparto sicurezza. La denominazione e l'origine stessa di questo Fondo dovevano dettare indicazioni ben precise, tanto che in sede di Commissione giustizia siamo arrivati ad una quarta formulazione dell'emendamento, che poi è stato votato. La Commissione giustizia ed anche la maggioranza avevano sostenuto e comunque almeno auspicato l'attribuzione di maggiori risorse al comparto della giustizia e contemporaneamente anche a quello della sicurezza. di fronte ad un taglio, ad una modifica normativa che riguarda il Fondo unico giustizia, e questo al di là di tutte le parole e di tutte le promesse che questo Governo di destra e questa maggioranza continuano a fare in materia di giustizia e di sicurezza.

che il sistema giustizia va completamente riformato; nel frattempo, al di là delle parole, non c'è alcun segno positivo in tal senso. Dico questo perché all'interno di questa norma, sulla quale viene posta la fiducia anche per smentire la propria maggioranza su questo punto, le risorse destinate al settore giustizia, e insieme anche al comparto sicurezza, vengono tagliate ancora una volta. ma anche ai nostri rappresentanti delle forze dell'ordine, agli operatori del sistema giustizia e del comparto sicurezza, che tutti i giorni lavorano sul territorio e sulle strade, che tutti i giorni combattono la criminalità e che tutti i giorni vengono a chiedere a questo Governo e a questa maggioranza di destra di far seguire alle parole i fatti. Ci troviamo di fronte invece all'insieme di tutti i sindacati di polizia e di tutti i rappresentanti della magistratura, che parlano di un fallimento e di un tradimento della politica di sicurezza di questo Governo. di un tradimento della politica di sicurezza di questo Governo. Il discorso è analogo rispetto al settore giustizia. Riteniamo che questa imposizione del voto di fiducia, che rientra sicuramente nelle facoltà

a voi di destra della sicurezza e della giustizia non vi interessa nulla; a voi interessa soltanto parlare, infinocchiare i vostri elettori e far credere al Paese

Altro che milleproroghe! In questo testo vi sono delle autentiche picconate al sistema giustizia, così come poc'anzi evidenziato dal collega Casson. Si era trovato il tesoretto, ossia quella massa di depositi mai utilizzati e risultanti dai libretti postali e bancari, oltre 2 miliardi di euro che erano destinati alla giustizia. dopo tanta enfasi, il Governo ha presentato un provvedimento per cui destinava soltanto il 30 per cento di quelle somme straordinarie - poi a regime ovviamente sono molto di meno

che «un cospicuo recupero di risorse finanziarie ci aspettiamo dal Fondo unico giustizia che abbiamo potenziato. Questo razionale sistema di utilizzo delle risorse finanziarie che l'attività giudiziaria produce da sé metterà finalmente a disposizione della giustizia notevoli risorse».

facendo salva questa risorsa straordinaria che finirà presto e, pertanto, a regime si andrà avanti con provvedimenti per i quali si prevede la rotazione; in sostanza,

che avviene attraverso un provvedimento al mese che demolisce pezzo per pezzo quello che faticosamente eravamo riusciti a costruire. Questa non è una proroga! provvedimento milleproroghe ci sono autentiche picconate. Non si vuole una giustizia che funzioni e non si vogliono dare risorse alla giustizia! Avete inserito un ulteriore intervento demolitore: avete demolito la Cassa delle ammende che aveva una specifica finalità, finanziare i programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore delle famiglie di detenuti ed internati nonché i programmi che tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione. Questa è tuttora la Cassa delle ammende. Con il vostro provvedimento, invece, inserite tra le finalità della Cassa delle ammende il finanziamento di progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Volete, quindi, costruire le carceri con la Cassa delle ammende: è la demolizione di un istituto che esiste dal 1932 con specifiche finalità!

Questo è un Governo che porterà al disastro il sistema Italia, perché non ha idee, non ha progetti, fa solo proclami e *spot*. Ancora ieri sera il Ministro della giustizia pontificava nelle reti televisive, parlando di giustizia di avanguardia, di interventi

avete inserito la norma sui processi agli immigrati, che costeranno 400 milioni di euro, per condannare gli immigrati a rimanere nella propria abitazione il sabato e la domenica per un massimo di quarantacinque giorni. Di fronte alle vostre ridicole soluzioni

colleghi, esponenti del Governo, questo ennesimo voto di fiducia avviene in un Senato dove vi è una maggioranza molto larga - e, mi pare, anche molto assente - e all'apparenza non trova spiegazione. Sicuramente vi sono problemi interni alla maggioranza, c'è incapacità e confusione nel governare; questo decreto milleproroghe ne è ulteriore conferma. Ma c'è anche una volontà ormai evidente di rendere il Parlamento un semplice luogo di ratifica delle decisioni del Governo. Con queste pratiche si attacca ulteriormente la Costituzione. Nello zibaldone - mi scuserà Leopardi per la citazione - di questo decreto-legge ci sono molti vuoti sul tema del lavoro e alcuni pessimi interventi sul medesimo tema. Molti vuoti: nonostante si cerchi di distogliere l'attenzione sulla crisi economica e del lavoro, la cassa integrazione aumenta e i provvedimenti, anche in questo decreto, sono insufficienti. La disoccupazione aumenta di due punti e non c'è nulla per i disoccupati. Di precari non se ne parla (anzi, questo decreto ne crea altri); molti di loro non hanno più il lavoro. Quando c'è un'emergenza si devono usare tutti gli strumenti: anche questo disegno di legge poteva servire a dare qualche risposta alle sofferenze del mondo del lavoro. Non illudetevi, non basta fomentare la paura e l'odio verso gli immigrati, scatenare guerre tra poveri, per risolvere i problemi di tante lavoratrici e lavoratori. La materialità e la crudezza della crisi renderanno evidenti le vostre inefficienze e i vostri errori. E non serve mettere mano, come state facendo, a leggi che restringono il diritto costituzionale allo sciopero. Uno dei primi deputati socialisti all'inizio del Novecento, Andrea Costa,

Era un emendamento della Lega (e mi addolora che rechi la firma di una sindacalista), approvato in Commissione affari costituzionali, che toglieva nei luoghi di lavoro con meno di 15 dipendenti i rappresentanti dei lavoratori

e le mansioni di questi rappresentanti erano e sono la priorità e la strada da seguire; formazione e prevenzione sono infatti le loro mansioni. Sono le solite scelte di questo Governo. Alla piccola impresa serve credito, innovazione, sostegno economico, non togliere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Poi c'è l'articolo 32, che proroga alcune norme sulla sicurezza contenute nel testo unico: è un segnale pessimo, così come sarebbe un pessimo segnale la modifica del testo unico prima ancora di averlo applicato. Ogni giorno in questo Paese muoiono dei lavoratori. La grave crisi di questi mesi accentuerà ancora di più il rischio di incidenti nei luoghi di lavoro. La concorrenza al ribasso, specialmente per le piccole e le piccolissime aziende, porterà ad un ulteriore decremento delle tutele per i lavoratori. La guerra tra poveri si giocherà anche, purtroppo, sui costi della sicurezza. In questo senso il Parlamento ha oggi una grave responsabilità: non inviamo messaggi ambigui, non si approfitti della crisi per passare sopra ai diritti e alla salute dei lavoratori. La sicurezza, la salute dei lavoratori, la lotta contro i morti sul lavoro sono una priorità per il Partito Democratico, sono una priorità tutti i giorni e non solo nel giorno del lutto a seguito delle grandi tragedie, perché tutti i giorni ci sono lavoratori che escono di casa e non ne fanno ritorno. Il testo unico si applica, non si cambia. Anche per queste ragioni voteremo no a questo disegno di legge.

ancora una volta prendiamo atto dell'ennesima fiducia che il Governo pone per l'approvazione rituale e stanca ad un atto come il milleproroghe, che si ripropone uguale a sé stesso nella forma, nella liturgia dell'*iter* d'approvazione e perfino nella ritualità della metodologia con cui si consumano vecchi e nuovi strappi all'ordinarietà e alla consuetudine istituzionale. Per carità, come veniva detto da un collega della maggioranza, niente di nuovo e scandaloso, se non se non fosse per l'insopportabilità di alcune circostanze che rendono questa situazione particolarmente odiosa, a partire proprio dal contesto politico in cui si consuma, immediatamente dopo uno dei peggiori spettacoli che quest'Aula abbia dato di sé agli occhi mediatici del Paese per volgarità e violenza verbale, consumato in un clima di furore ideologico degno di altri tempi, uno spettacolo da baraccone organizzato nella convulsione e nella compressione di tempi televisivi funzionali più a quello scopo che all'obiettivo del provvedimento: ha mandato in scena l'imprevisto dramma del fine vita di Eluana in cui tutti noi inevitabilmente ci siamo, almeno per un attimo, impersonati, forse più nell'icona della giovane sorridente che nel simulacro del corpo che giaceva in quel letto. Ma il Parlamento in quella circostanza era chiamato a fare presto e bene per salvare - veniva detto - quella vita e in futuro molte altre come quella. La morte sopraggiunta di Eluana ha reso vano tutto quell'affanno compulsivo, ma forse non è stata inutile se - come ci siamo impegnati tra noi - in un tempo più ragionevole (poche settimane appena), riusciremo a definire almeno una cornice normativa minima in cui inquadrare situazioni estremamente delicate e complesse come quella in cui si è consumata l'intera vicenda degli Englaro e dimostrare la volontà di recuperare davvero la nostra credibilità agli occhi dei cittadini. Forse l'auspicio anche che da un male (la morte di Eluana, il pessimo spettacolo dato, le tensioni che si sono consumate intorno a quel dramma) possa nascere anche un bene, un minimo di certezza normativa che possa aiutare chi si trova a vivere queste non auspicabili circostanze può non essere una pia illusione. Oggi invece, passata la tempesta mediatica, è come se tornassimo alla peggiore bonaccia, offrendo per il lato opposto il nostro più deteriore spettacolo, consumato senza attenzione pubblica, con un'Aula -viene ricordato - pressoché deserta e con i pensieri della maggior parte di noi rivolti altrove, come se nascondessimo a noi stessi che proprio in questa settimana sono andate paradossalmente in scena le due facce singolari ed opposte della stessa medaglia, quella cioè di un Parlamento che rischia ormai di essere il simulacro agonizzante di sé stesso, capace ormai solo di qualche sussulto retorico quando gli vengono accesi i riflettori e poco più. Presidente e colleghi, soprattutto della maggioranza, portiamo una bella responsabilità su di noi: la responsabilità di contrastare la percezione ormai prevalente nell'opinione pubblica della nostra (intendo come Parlamento e come singoli parlamentari) inutilità. Paradossalmente è proprio da atti apparentemente insignificanti come questo, dal modo in cui si affrontano e da quello in cui si risolvono e si concludono che si contribuisce ad avvalorare proprio quella percezione dalla quale noi per primi dovremmo rifuggire. Non so quanto serva ogni volta ricordarvi che i vostri numeri, colleghi della maggioranza, dovrebbero consentirvi agevolmente altri e più consoni comportamenti. Perfino il richiamo alla vostra intelligenza, non dico alla vostra sensibilità, ma almeno all'orgoglio istituzionale, dovrebbe quantomeno indurvi ad un atteggiamento teso ad una maggiore salvaguardia delle prerogative proprie delle Aule parlamentari. Un Parlamento invece che sembra ridotto, e ve lo ripeteremo ogni volta che lo mortificherete o acconsentirete a mortificarlo, ad un organo di ratifica in cui si agisce per decretazione, spesso accampando motivi di necessità ed urgenza per poi tentare, nell'*iter* di approvazione, qualche assalto o incursione alla riforma surrettizia degli ordinamenti. Sul provvedimento, purtroppo, poco o niente da dire, se non, lo ripeto, il protrarsi stanco di scadenze rimandate a cui Governo o Parlamento non sono stati in grado di adempiere, intercalate da provvedimenti che in molti casi si rivelano opposti rispetto a come si definiscono e altri che avrebbero richiesto un momento maggiore di confronto. È il caso dell'emendamento sulle concessioni autostradali, che ripristina *sic et simpliciter* la situazione *ex ante* il famoso articolo 12 introdotto dal ministro Di Pietro, senza lo straccio di una riflessione o di un confronto di merito, come invece avrebbe meritato. È il caso anche di provvedimenti che, anziché semplificare, continuano a complicare la vita ai cittadini e alle imprese, rendendoci ogni giorno più distanti e incomprensibili da loro. Tutto ciò, a mio avviso, ma - credo - non solo mio avviso, costituisce la plastica rappresentazione di un Governo immobile che, anziché affrontare, si nasconde dietro questa crisi che al contempo è sempre più, non solo economica, ma anche di valori e di responsabilità.

nel corso del dibattito sul decreto milleproroghe noi dell'Italia dei Valori avevamo posto in evidenza

alla prassi adottata e non penso al modello delle milleproroghe nei confronti del quale l'attuale maggioranza, quando era opposizione,

sono un segnale, una spia, di incapacità della pubblica amministrazione di far fronte ai propri adempimenti. Ma al di là della tesi che fu sostenuta all'epoca dal centrodestra, torniamo alla

Penso al rinvio della normativa sugli infortuni sul lavoro. Siamo stati attenti ascoltatori della lezione del senatore Pera sui principi sui principi e sui diritti inviolabili della Costituzione. Crediamo che per ogni lavoratore e per ogni cittadino italiano e non italiano la sicurezza sul lavoro sia anch'essa un diritto inviolabile. L'Italia

tema. Avevamo criticato poi la norma che rinviava ulteriormente l'esame del problema relativo all'IRAP e alle tasse automobilistiche. Non ci eravamo scandalizzati del fatto che quell'ulteriore rinvio avrebbe determinato una ennesima mancanza di attuazione delle promesse elettorali che il presidente Berlusconi aveva fatto durante la campagna elettorale, nel corso della quale aveva dichiarato a tutti gli italiani che avrebbe abolito le tasse automobilistiche, ma con questo decreto milleproroghe ne rinviamo l'esame e, quindi, le confermiamo.

per poi scoprire nel mese di dicembre che dell'elenco ISTAT (che comprende oltre 340 enti), con tutti i distinguo, le proroghe e le deroghe, si era arrivati a individuare nove enti anche questi nove enti, nonostante i grandi annunci roboanti dei Ministri del Governo Berlusconi, alla fine sono stati salvati.

una terza criticità, che è stata rilevata in maniera competente e sobria da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, e che è ravvisabile nella trasformazione del Parlamento in una fabbrica passacarte: questa è la fotografia dell'attuale Parlamento italiano. Una fabbrica passacarte che, però, ha dei costi ha dei costi e non soltanto quelli esclusivamente tecnici e procedurali legati alla stampa delle migliaia e migliaia di carte che si ripetono e si aggiungono: ha dei costi che sono stati rilevati in maniera estremamente competente dalla stessa Corte dei conti. Chi ha avuto la pazienza di leggere la relazione annuale della Corte dei conti sulle

che, essendo anche segretario del Sindacato padano, io possa essere favorevole all'abolizione della figura che deve tutelare e segnalare all'interno delle aziende quello che non funziona.

sappiamo come finisce: escono gli articoli sui giornali, però in quelle aziende si continua a lavorare come prima. Figuriamoci se potevo essere d'accordo con un emendamento del genere! Ho chiesto con forza che tale emendamento venisse ritirato

cari colleghi, siamo davvero di fronte ad un provvedimento rituale - è stato sottolineato da più interventi - che stancamente ogni anno viene riproposto. La ritualità, però, trova un limite nei contenuti e nelle modalità stesse con cui questo provvedimento di anno in anno viene riproposto di fronte alle Camere. Quest'anno esso è indubbiamente più denso che mai di proroghe, di prolungamenti di termini, ma anche di piccoli ma significativi elementi che vanno oltre l'elemento caratterizzante della proroga dei termini.

qui ricordato da diversi colleghi (dai colleghi Vita, Ceccanti ed altri), sull'editoria, sull'ambiente, su alcuni aspetti che riguardano la fiscalità e così via; che abbiamo contribuito a migliorare togliendo norme che non condividevamo e che avrebbero prodotto danni: penso al rinvio del riordino degli enti di ricerca e al tema della giustizia amministrativa. Avremmo voluto contribuire a migliorarlo in Aula, assieme alla maggioranza, se non fosse intervenuto questo voto di fiducia capestro che toglie ogni possibilità di confronto: lo toglie a noi, lo toglie anche alla stessa maggioranza, come qui è stato plasticamente evidenziato dall'intervento della senatrice Mauro. Non si è potuto migliorare questo provvedimento nei contenuti. Penso al tema dell'agricoltura, su cui si è soffermato il collega Andria; un tema ed un settore che non è stato per nulla interessato dagli interventi anticrisi che il Governo ha promosso nelle scorse settimane e che avrebbe potuto trovare in questo provvedimento, con il consenso di tutti, alcune modalità anche di alleviamento di una serie di vincoli, a cominciare dal contenzioso previdenziale, che stanno stringendo molte aziende in tutto il Paese. Infine, non abbiamo potuto migliorare questo provvedimento su uno degli elementi forse più significativi: l'ulteriore rinvio della norma della cosiddetta *class action*. Voglio soffermarmi brevemente su questo aspetto perché mi sembra uno degli elementi più significativi. Si rinvia ulteriormente a giugno l'entrata in vigore di questa norma con un decreto-legge su cui viene posta la fiducia. È un segno ulteriore, accanto a molti altri, della politica di questo Governo, che intende contrastare nei fatti, come sta facendo, una norma moderna, di civiltà economica, prima ancora che giuridica; una norma che ha messo al centro della legislazione del nostro Paese, nel rapporto tra i grandi gruppi economici ed i cittadini, una nuova figura, il cittadino consumatore, che ha bisogno di tutele adeguate e di salvaguardia: un nuovo protagonista nella vita nel Paese. l'ampio dibattito svoltosi nelle Aule parlamentari nella precedente legislatura sulle cosiddette leggi Bersani, al cui interno la norma della *class action* ha trovato spazio importante e significativo. non si tratta solamente e semplicemente di non lasciare impuniti i responsabili di disastri finanziari ed economici che in questo Paese, negli ultimi anni - consentitemi di dire - l'hanno fatta spesso franca, di chi ha fatto un cattivo uso del mercato. Si tratta di questo, certo, ma soprattutto di stimolare una maggiore e migliore qualità nel rapporto tra i cittadini ed i grandi gruppi economici; una migliore qualità dei servizi. Insomma, non è un caso se gli indici sulla libertà economica, appena pubblicati qualche giorno da autorevoli osservatori internazionali, consegnano all'Italia un disonorevole sessantaseiesimo posto, agli ultimi posti, dopo Paesi lontani per qualità della democrazia, per storia e potenzialità economica; siamo dopo Cipro, dopo l'Albania, dopo il Botswana: lascio i commenti a chi vorrà. Di questo stiamo parlando, cioè di una nuova epoca di rapporti tra il sistema economico, il mercato, il cittadino consumatore. Ebbene, vi approverete tra qualche istante una ulteriore proroga di questa norma. Vi solleciteremo nelle prossime settimane affinché il 30 giugno, data di scadenza di questa ulteriore proroga, non ve ne siano di ulteriori. Lo dobbiamo ai cittadini del nostro Paese, ai cittadini consumatori, a tutti noi. Lo dobbiamo anche al sistema delle imprese, quello sano, di questo Paese che non ha alcuna paura e timore di queste norme. Ancora, Presidente, avremmo voluto migliorare questo provvedimento, ma non è stato possibile perché il Governo ha portato qui un decreto‑legge con tempi contingentati ed ha posto sullo stesso, per l'ennesima volta, la questione di fiducia; insieme, decreto‑legge e questione di fiducia. Probabilmente lo fate, signori del Governo e della maggioranza, per tenere insieme una coalizione che magari non ha le stesse idee su tante questioni. lo fate per impedire un confronto che avrebbe portato a valorizzare il ruolo di queste Aule e anche della dialettica parlamentare. Lo fate probabilmente perché voi stessi avete ingolfato le Camere e il Parlamento presentando solo con decreti‑legge, che, avendo una scadenza precisa, hanno bisogno di essere esaminati e votati in tempi ristretti. Avete ingolfato il Parlamento comprimendone il ruolo sacro. Siamo di fronte - è un tema su

a spostare sempre più la funzione legislativa dalla sua sede naturale e costituzionale, dalle Aule del Parlamento, ad un'altra sede, un Parlamento ridotto a votificio. Si tende a spostare questa funzione sacra ad un'altra sede, a quella della funzione esecutiva, che è propria del Governo. C'è financo chi lo teorizza: il presidente Berlusconi ha affermato che l'unico modo di governare è decretare d'urgenza, salvo poi

in questi mesi solo una legge di iniziativa parlamentare ha trovato l'approvazione delle Aule del Parlamento del nostro Paese. Su tale aspetto dovremmo quindi riflettere affinché tale processo di spostamento progressivo della funzione legislativa dal Parlamento al Governo venga bloccato e vengano bloccate le mire di qualcuno (a cominciare dal Presidente del Consiglio, che non se ne fa ombra di dichiararlo) a portare avanti questo disegno delittuoso della Carta costituzionale. Avete decretato in questi mesi su tutto, salvo poi aggiungere ai decreti-legge la fiducia;

di una sorta di disagio istituzionale di cui in quest'Aula, tutti insieme, dovremo farci carico. Per queste motivazioni, caro Presidente, il voto del Partito Democratico sarà contrario a tale provvedimento ed alla fiducia richiesta.

al collega, il nostro Gruppo voterà a favore, come dirà il collega che farà la dichiarazione di voto, per una serie di argomenti che sono opposti a quelli che finora abbiamo ascoltato. Fra i molti temi che questo decreto contiene, ne distinguo uno, che consente di recuperare una situazione di svantaggio e di disagio causata da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che impone il pagamento dell'ICI anche per i fabbricati rurali. Ne hanno già parlato alcuni colleghi, ma nessuno qui ha ricordato che già prima dell'iniqua sentenza del Consiglio di Stato era stata proposta un'iniziativa legislativa dall'allora ministro Visco del Governo Prodi che che stabiliva esattamente la stessa cosa. Con questo decreto-legge rimediamo a quell'atto che riteniamo ingiusto e proponiamo di perequare in maniera positiva per gli agricoltori, soprattutto quelli di montagna. Questa esenzione dell'ICI tocca non soltanto fabbricati agricoli così definiti, ma anche quelli che non danno più reddito, che non sono essenziali per l'esercizio dell'attività agricola primaria, ma che sono, viceversa, un onere, un peso, un costo netto per il proprietario. un contrasto anche con il dettato della legge n. 212 del 2000 e del decreto legislativo n. 504 del 1992.

dell'applicazione dell'ICI a certi fabbricati rurali e, in particolare, a edifici che in montagna nemmeno potrebbero essere definiti tali. Per le zone di montagna a soccorrere questo tipo di iniziativa c'è anche la legge n. 97 del 1994 che è in attesa di una revisione; è già stato depositato un testo firmato da oltre 60 senatori di questa legislatura e che attende di essere incardinato. legge suggerisce l'esenzione dell'ICI per quei fabbricati che contribuiscono a mantenere vivo il patrimonio naturale e paesaggistico di una località di montagna, oltre ad essere complementari e necessari ad un'attività professionale agricola. A sostegno di questa tesi, infine, c'è anche il regolamento comunitario n. 1260 del 1999, il quale riconosce

carenza di servizi e scarsi redditi da attività agricole e per altri motivi che hanno contribuito a delineare la definizione di zona svantaggiata, oggi respinta da molte località di montagna, ma che esiste comunque nel frasario delle legislazioni L'esenzione dell'ICI non risolve certamente tutti i problemi che ho elencato, ma dà un segnale di attenzione importante a chi decide di continuare a vivere e a lavorare in tali condizioni certamente non vantaggiose. In realtà, lo svantaggio non è endemico, non è legato al territorio o provocato da questo, ma deriva dalla scarsa oculatezza dei legislatori e degli amministratori, in sostanza di coloro che devono applicare la legge.

Grazie, una specificità alla quale intendo richiamarmi in maniera molto insistente e convinta - servono come ricovero per attrezzi, piccoli fienili, attività forestali, ma talvolta anche per attività di ricreazione e di ritrovo. in molte località questi edifici sono soggetti a vincoli anche paesaggistici sui quali non possono intervenire, da parte del proprietario, anche se lo volesse, cambiamenti delle destinazioni d'uso nelle strutture sia esterne che interne. Ecco, in base a tutto quello che ho detto si crea una situazione davvero perniciosa per l'agricoltore o l'allevatore di montagna che si trova ad essere proprietario di questi fabbricati. Innanzitutto non gli

né ha alcuna possibilità di alienarli, ad esempio, al cittadino di passaggio che potrebbe ricavarne un rifugio per le sue gite o magari per un soggiorno turistico estivo. però, il proprietario di questi edifici non provvedere alla loro conservazione, che richiede - è inevitabile - costi, in quanto, se non fossero conservati e accuditi, finirebbero per crollare, il che diventerebbe una colpa. Quindi, non ha redditi,

passa questo decreto-legge - come ci auguriamo noi tutti, almeno da questa parte - questo tipo di balzello non ci sarebbe più. Di qui la proposta di esenzione per gli agricoltori a pieno titolo: per essere chiari fino in fondo, è lapalissiano che se questi edifici dovessero essere autorizzati a cambiamenti d'uso o passaggi di proprietà, per diventare per esempio case per le vacanze, in quel caso legittimamente tutti sarebbero tenuti a pagare l'ICI, ma certamente non il proprietario originario.

essa va a toccare un equilibrio socio-economico già di per sé molto fragile. Soprattutto, questa crisi va ad incidere sul reddito di professionalità molto empiriche, a volte anche precarie e multifunzionali;

chiudere questa bombola, essenziale per la continuità delle attività professionali in montagna e nelle zone rurali svantaggiate, quindi anche per la vita della gente che crede in questo impegno e in questa professione. *(Applausi

Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il provvedimento sul quale l'Esecutivo ha posto la questione di fiducia, il cosiddetto milleproroghe, rappresenta certamente un'anomalia che sistematicamente si rinnova, trasformando l'eccezione in sistema: di semestre in semestre, da Governo a Governo, l'eccezione diventa la regola che in qualche modo consente allo Stato e all'amministrazione di tirare a campare. I provvedimenti che prorogano i termini previsti per l'attuazione di provvedimenti legislativi non sono certamente un'invenzione di questo Governo, ma ci auguriamo che, invece, merito di quest'ultimo sia interrompere tale prassi negativa, scegliendo e razionalizzando. Allo stato delle cose, però, un tale provvedimento rappresenta, almeno nel suo complesso, niente di più che un atto dovuto e un indispensabile strumento, rispetto al quale appaiono prive di senso molte speculazioni politiche. È per tale ragione che in questa occasione noi del Movimento per l'Autonomia non abbiamo particolare difficoltà a dare la nostra fiducia al Governo. Quale forza politica della maggioranza parlamentare che sostiene con lealtà l'azione dell'Esecutivo, non possiamo però in questa sede non ribadire con forza la nostra posizione. Pur non avendo infatti i numeri per influire in maniera significativa sulle priorità del Governo, anche rivolgendoci direttamente al Presidente del Consiglio, ancora una volta ribadire con molta nettezza che la politica governativa non sta rappresentando sino ad ora il giusto riconoscimento per i tanti elettori del Mezzogiorno, che con il proprio voto hanno consentito la vittoria elettorale alle elezioni politiche dello scorso anno. Sono ormai trascorsi molti di più dei 100 giorni iniziali; siamo a dieci mesi e non c'è traccia, nei tanti provvedimenti varati dall'Esecutivo, di misure veramente significative in favore del Sud. Anzi, c'è il rischio fondato che su alcune questioni fondamentali si siano fatti passi indietro. In particolare, nell'azione del Governo ancora non vi è traccia di quell'impegno previsto al quinto punto del programma di Governo: politiche che consentano il superamento del divario tra Nord e Sud. C'era anche questo nel programma elettorale: ridurre, ed in prospettiva annullare, il divario tra Nord e Sud; chiedere ad un grande Paese come il nostro di fare quello che la Germania ha fatto in pochi anni nei confronti dei territori che costituivano l'ex Germania dell'Est. È questo l'impegno che è stato preso alle elezioni ed è questo che giustifica ancora la presenza del Movimento per l'Autonomia nella coalizione di Governo. Non nascondiamo la nostra forte preoccupazione, ed in parte la nostra delusione, perché ancora poco di significativo, come detto, in questa direzione è stato attuato. Il Movimento per l'Autonomia, attraverso i suoi due senatori, otto deputati e i suoi due due Sottosegretari, non ha - lo ribadisco - i numeri per determinare una sterzata in favore del Mezzogiorno, sia in termini di stanziamenti finanziari per le opere pubbliche sia in termini di politiche fiscali che rilancino gli investimenti privati; si deve limitare a chiedere con forza all'Esecutivo il rispetto degli impegni presi con gli elettori, senza fare a meno di osservare che le parole impegnative di qualche settimana fa del ministro dell'economia Giulio Tremonti («dobbiamo impegnarci tutti sulla grande questione dell'Italia che è il Mezzogiorno») si traducano in Consiglio dei Ministri in atti concreti. Vorrei dire al Ministro dell'economia che è vero che uno dei grandi problemi per il Sud è stata proprio la sua classe dirigente, che ha talvolta indegnamente rappresentato in Italia e all'estero il Mezzogiorno e l'Italia intera. È anche troppo comodo però non prendere atto dal fatto che una parte della classe politica del Mezzogiorno sta iniziando concretamente, con atti di governo, con riforme coraggiose, e spesso solitarie, a riscattare un'immagine di un Sud sprecone e più o meno intriso di una cultura mafiosa, che favorisce interessi privati a scapito della comunità. In Sicilia, il presidente della Regione Raffaele Lombardo, senza clamori e con sobrietà, come gli è consueto, sta rappresentando una classe politica che ha deciso di fare della responsabilità e del contrasto alla criminalità mafiosa la bussola per la concreta azione di Governo. Questa classe dirigente che il Movimento per l'Autonomia - per carità, anche insieme ad altre forze - si sforza di rappresentare in Sicilia, anche nelle altre Regioni del Mezzogiorno, chiede al Governo di fare la sua parte, facendo, come in tanti molto più autorevoli di me da anni affermano, del Mezzogiorno una opportunità per l'intero Paese. Questo Esecutivo può avere il consenso e la determinazione per mettere in campo politiche economiche coraggiose che, anche facendo uso della leva fiscale, riescano, in questo periodo particolarmente difficile, a convogliare al Sud capitali e imprese. Grazie,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto che stiamo per approvare, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, e per il quale annuncio il voto contrario del Gruppo UDC, SVP e Autonomie, reca la proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative che riguardano diversi ambiti settoriali, tra cui difesa, pubblica amministrazione, lavoro, infrastrutture e trasporti, affari esteri, agricoltura, sviluppo economico, istruzione, beni culturali, ambiente, finanze e numerosi altri ancora. Prima di entrare nel merito del provvedimento, vorrei far osservare che, nonostante i ripetuti richiami ad una maggiore chiarezza dei testi normativi da parte del Governo, numerosi articoli del decreto-legge non indicano esplicitamente il contenuto delle disposizioni a cui si riferiscono. (e questo aspetto è già stato oggetto di discussione in Commissione), molte disposizioni mancano del requisito di urgenza e molte altre trattano le materie più svariate e, pertanto, risultano talmente eterogenee che poco attengono a proroghe di termini. Relativamente al primo aspetto, in sede d'esame del provvedimento in prima Commissione, sono state giudicate ampiamente insufficienti le motivazioni di urgenza addotte dal Governo per il differimento dell'entrata in vigore di alcune norme, ed in particolare quelle relative alla *class action*, quelle relative all'entrata in vigore delle limitazioni alla guida di veicoli per i neopatentati, nonché quelle relative ai termini di applicazione delle disposizioni in materia di comunicazione

quelle che attribuiscono nuovi ed ulteriori poteri al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di bilancio dello Stato. Infatti, assai singolari sono le disposizioni concernenti l'emissione dei titoli pubblici e, in particolare, i poteri attribuiti in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione, come ho già accennato, il Governo ha presentato diversi emendamenti non attinenti a proroghe di termini tra questi, voglio citare l'emendamento relativo al potenziamento delle infrastrutture carcerarie. In definitiva, mi sembra che la proroga ripetuta di termini non faccia altro che testimoniare l'inadempienza delle amministrazioni: in tal modo si accresce l'incertezza degli operatori e dei destinatari circa la necessità di adeguarsi alle leggi. Inoltre, il continuo differimento si traduce in una nuova forma di intervento legislativo. Per quanto riguarda il merito, la non tempestiva soppressione di enti inutili comporta oneri finanziari che sembrano ignorati dalla relazione tecnica, mentre l'ulteriore differimento della *class action* si configura come una sostanziale violazione della legge da parte del Governo. Il decreto-legge in esame non reca alcuna misura anticrisi per sostenere i redditi più bassi e contrastare la disoccupazione, ma attraverso attraverso misure quali la proroga dell'IRAP e delle tasse automobilistiche aumenta le incertezze degli operatori e contravviene all'impegno del Governo di ridurre la pressione fiscale. Oltre ad essere disomogeneo, il decreto-legge è contraddittorio rispetto alla stabilizzazione dei precari nelle amministrazioni pubbliche: infatti, si consente ai Ministeri, dopo aver ridotto gli organici, di prorogare i contratti di lavoro a termine. È evidente quindi - e concludo - che la necessità di intervenire con numerose proroghe dipende dalla mancata capacità di indicare termini adeguati in sede di produzione legislativa e amministrativa. Inoltre, mentre mentre può comprendersi l'esigenza tecnica di prorogare i termini di alcune norme, si dovrebbe adottare maggiore cautela quando si tratta dell'entrata in vigore di leggi: in tal caso il differimento si configura come una configura come una forma impropria di tecnica legislativa. Per queste ragioni dichiaro che il mio Gruppo non appoggerà il voto di fiducia e, quindi, esprimerà

Prego, senatore Pardi. lodi sperticate di una finanziaria rivoluzionaria, che avrebbe risolto i problemi dello Stato per tre anni; invece da allora, dall'inizio della legislatura, si sono succeduti

su circa 45 giorni di possibile dibattito, sul milleproroghe si è discusso, in modo scarso, per soli due giorni (naturalmente non per l'intera giornata). Questo la dice lunga sulla possibilità del Parlamento di discutere, criticare, emendare, migliorare provvedimenti di qualsiasi natura, soprattutto quelli di natura finanziaria, che sono alla base del nostro comune vivere.

Prima di tutto, bisogna osservare che in questo maxiemendamento sono entrati pezzi di provvedimento che non sono transitati in nessuna Commissione di merito; sono stati infilati senza che le Commissioni di merito, e tanto meno la Commissione bilancio, abbiano potuto discuterne. Poi c'è l'abominio giuridico della proroga dei termini. Oramai la proroga è diventata una forma normativa stabile e ordinaria, rafforzata - come si vede ancora oggi - dalla fiducia. All'interno di questi meccanismi entrano alcuni piccoli mostriciattoli. L'articolo 7-*bis*, ad esempio, anticipa l'entrata in vigore di alcune misure del cosiddetto disegno di legge Brunetta, che in realtà è ancora all'esame del Parlamento. infilano quindi dentro il maxiemendamento, con un atto forzoso, delle norme che sono in discussione nell'altro ramo del Parlamento. Ci si chiede se questo non dipenda da un'allergia del Governo al dibattito parlamentare. Evidentemente l'Esecutivo ritiene necessario far svicolare come serpi pezzi delle proprie intenzioni all'interno dei provvedimenti. curioso che, nell'anticipazione della crociata antifannulloni del ministro Brunetta, si trovi addirittura, all'articolo 10, una promozione di funzionari del Ministero degli affari esteri senza concorso: questa è la maniera migliore per dimostrare che noi invochiamo la meritocrazia e sottoponiamo a vaglio la promozione del nostro personale.

sono tutti particolari concordanti in un'unica direzione. Poi ci sono le prebende e gli ammiccamenti pre-elettorali: norme misteriose per gli agricoltori sardi. Sappiamo che il Presidente del Consiglio nell'ultimo mese, invece di guidare il Governo, ha essenzialmente fatto campagna elettorale in Sardegna, pare comprandosi l'ultima l'ultima televisione che c'era sul mercato, e ovviamente non ci si poteva che aspettare dei provvedimenti per gli agricoltori sardi. Poi c'è un favore al CONI, di dubbio un fatto umoristico: la liberalizzazione delle molestie telefoniche; inutilità) dovesse crescere, possono sfogarsi impunemente con le molestie telefoniche, da loro stessi organizzate.

Prima di tutto, il Parlamento è all'oscuro dei conti, perché manca la relazione sul secondo semestre; quindi noi ragioniamo su una cosa di cui non sappiamo niente.

modificare le suddette procedure al fine di rendere più efficiente il processo di vendita». Si sapeva che nella nostra società, per essere efficienti, bisogna cambiare le regole; ce lo ha insegnato il Presidente del Consiglio, che si è fatto le leggi *ad personam* per uscire dai processi, e questa è una piccola manifestazione vernacolare di questa vocazione.

immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico». Quale sia la tecnica scientifica per stabilire quantitativamente cosa sia un apprezzabile risultato economico il testo non ci dice, ma noi ne ricaviamo la sensazione che tutto l'insieme non può essere apprezzabile. Senatore Pardi, se lei tace noi ascoltiamo quello che dice il senatore La Torre.

danni inenarrabili e forse irrimediabili al recupero dei carcerati. La manovra fiscale e finanziaria aveva promesso procedure rigorose, norme anticrisi e una regola del risparmio. Qui invece si assiste ad una distribuzione e a una dissipazione che parte - lo ricordo - dalla voragine Alitalia, che sarà pagata dal contribuente italiano, e arriva ai fondi per l'Expo di Milano, fino alla contribuzione alle Regioni a statuto ordinario che confinano con l'Austria per l'acquisto di carburante. Si capisce la sottigliezza, ma in una situazione di questo tipo forse non ce n'era bisogno.

Ciò detto, la Lega Nord voterà la fiducia, non tanto perché ha trovato soddisfazioni particolari o perché siano state accolte chissà quali richieste: anzi, per dirla tutta, di richieste della Lega ne sono state accolte ben poche;

aumentare la quota di interessi deducibili, assolutamente importante ed utile adesso perché le nostre imprese soffrono in particolare nel settore del credito visto che le banche hanno stretto i cordoni della borsa; rimettere la possibilità degli ammortamenti anticipati,

Quindi è un cambiamento di rotta a 180 gradi rispetto ad un certo modo di agire (il milleproroghe di Prodi). Finalmente si premia, e si premiano i Comuni e gli enti locali che hanno operato bene e hanno rispettato i patti.

di poter investire, perché gli investimenti da parte dei Comuni rappresentano il primo volano dell'economia, il primo modo per rimettere veramente in circolo un po' di quattrini soprattutto a favore delle nostre aziende (è evidente a tutti che le asfaltature, almeno quelle, non si possono importare).

Abbiamo bisogno che queste piccole e medie imprese vengano aiutate sotto due aspetti. In proposito, ricordiamo che la Lega ha già ottenuto (ed è importante) la revisione congiunturale degli studi di settore, che dovrà concludersi a breve, entro marzo, e dare sicurezza e certezza alle piccole imprese che stanno

il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo provvedimento con grande convinzione, non tanto per il contenuto specifico, su cui ci sono molte riserve che sono già state illustrate, ma per la grave, ennesima forzatura. Al riguardo svilupperò tre punti. Primo punto: la questione dei maxiemendamenti associati alle fiducie.

Ma esiste anche un'Aula di questo Senato ed esiste anche la Camera dei deputati presso cui vi accingete, evidentemente, a porre di nuovo la fiducia. Lo sappiamo tutti: avremmo potuto finire i lavori anche prima della fiducia e senza la fiducia. I maxiemendamenti servono a proteggersi dalla propria maggioranza. Voi rivelate di aver paura della vostra maggioranza. L'avete compressa con i decreti, con la finanziaria "snella", ma chi è troppo compresso finisce poi per esplodere. Avremmo finito prima e, forse, avremmo finito diversamente. Non so se meglio o peggio, però potevamo decidere in maggiore libertà. maggiore libertà. Immagino già la risposta, che vedo riflessa nell'espressione del ministro Vito: chi è senza peccato scagli la prima pietra; non avete inventato voi i maxiemendamenti? Di peccati ne abbiamo tanti e non solo negli ultimi due anni, è vero. Ma partiamo anzitutto dai numeri, che non sono uguali: voi avete proposto sei maxiemendamenti, con una media di 0,7 al mese;

C'è poi una differenza qualitativa rilevante: noi avevamo una maggioranza di micropartiti. Per i nostri peccati abbiamo già pagato alle elezioni decidendo di andare con una linea diversa, non più di coalizioni litigiose. Abbiamo voluto aprire una nuova stagione, la stagione dei maxigruppi, non quella dei maxiemendamenti, mentre voi continuate invece a proporre i maxiemendamenti in presenza di maxigruppi: non è la stessa cosa. riferimento alla questione della decretazione d'urgenza. Avevamo capito, all'inizio della legislatura, che volessimo tutti ridurre al minimo l'uso abnorme di questo strumento, anche tenendo conto degli orientamenti restrittivi della Corte costituzionale. Richiamo in ultimo la sentenza n. 128 del 2008, la quale ci ha ricordato che la legge di conversione non funziona da sanatoria per eventuali difetti dei decreti originari.

bensì di una precisa linea di rispetto della *ratio* sostanziale che ha sostenuto la scelta del legislatore costituente: quella di attribuire al Governo un potere legislativo del tutto eccezionale» - sottolineo, del tutto eccezionale «assoggettato alla conversione dell'atto normativo in legge». Per inciso, non risultano smentite del Presidente del Consiglio a sue dichiarazioni attribuitegli da un articolo del quotidiano "LaStampa" di oggi in cui interviene sui giudici da nominare alla Corte costituzionale e su chi sia più auspicabile che svolga la funzione di presidente della Corte stessa. Forse qualcuno dovrebbe ricordargli che questi poteri non sono nella sua disponibilità.

ad una di 3,7 al mese. I numeri non sono gli stessi. E avevamo ragionato di opportune modifiche regolamentari per applicare la Costituzione. Sappiamo, infatti, che l'articolo 72 della Costituzione, che indica la via di una corsia preferenziale per la rapida votazione di leggi, senza comprimere a dismisura i tempi di una ragionevole istruttoria legislativa, è stato sostanzialmente disatteso e per questo il presidente Flick, nel medesimo intervento del 28 gennaio, ricorda che «soltanto le forze politiche in Parlamento possono elaborare - attraverso correttivi regolamentari meccanismi destinati ad accelerare l'*iter*di formazione delle leggi». Noi restiamo a quell'approccio ragionevole, dentro la Costituzione, per applicare la Costituzione Invece, il Presidente del Consiglio sembra ispirarsi in questi giorni ad un'altra Costituzione. Proprio lui, che ha accusato la nostra di essere filosovietica, ignora evidentemente che la Costituzione di Stalin del 1936 (ho qui con me il testo prevedeva decreti del Governo senza il controllo di una figura di Capo dello stato. Si travolgerebbe così, con l'idea esposta più volte in questi giorni dei decreti senza controllo presidenziale come via normale di decisione, non solo la nostra Costituzione ma il patrimonio profondo del costituzionalismo democratico. L'articolo 16 della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 ricordava che ogni società nella quale non vi è garanzia dei diritti e separazione dei poteri non ha costituzione. Il legame tra garanzia dei diritti e separazione dei poteri è indissolubile: non sono principi negoziabili. In terzo luogo, la questione democratica e il fastidio per i vincoli. Il presidente Pera l'altro giorno ci ha proposto alcune interpretazioni suggestive ma infondate, e per certi versi pericolose, dell'articolo 2 della Costituzione. La clausola di apertura a diritti non scritti, contenuta all'articolo 2, per cui i diritti vengono prima dello Stato, non significa che i diritti che vengono prima dello Stato possano essere interpretati contro la Costituzione e comunque non vi sono, al di fuori dei poteri previsti dalla Costituzione, interpreti univoci e astorici. Fornirò al presidente Pera, dal "Commentario alla Costituzione" Zanichelli, il commento del professor Barbera all'articolo 2 della Costituzione. Dice il professor Barbera: «Quale che sia l'arricchimento che può provenire dal richiamo di un ordine naturale e razionale, sia pure inquadrato in una dinamica storica, non può non rinvenirsi in esso un grosso rischio: di considerare presupposto dell'ordinamento ciò che invece ne è il fine. Il libero sviluppo della persona è un "compito" da realizzare e non solo un "dato" da rispettare(...). Il problema diventa quello di modellare l'organizzazione del potere pubblico non solo in funzione della garanzia dei valori della persona (come nelle vecchie teorie giusnaturalistiche e come in molte di quelle moderne), Negri)*. Per di più, vorrei dire che neanche la Chiesa cattolica, dopo il Concilio Vaticano II e in particolar modo dopo la «*Dignitatis Humanae*» e la «*Gaudium et Spes*», interpreta quel richiamo al diritto naturale nel senso ingenuo fornito dal senatore Pera, quale vorrei ricordare quello che, per l'appunto, diceva il cardinale Joseph Ratzinger nel dialogo con Jürgen Habermass. Dice il cardinale Ratzinger: «Il diritto naturale è rimasto, soprattutto nella Chiesa cattolica, la figura argomentativa con cui essa richiama alla ragione comune nel dialogo con le società laiche e con le altre comunità di fede e con cui ricerca i fondamenti di una comprensione attraverso i principi etici del diritto in una società laica e pluralista. Ma questo strumento» - attenzione - attenzione - «è purtroppo diventato inefficace, e non vorrei basarmi su di esso in questo intervento. Il concetto del diritto di natura presuppone un'idea di natura in cui natura e ragione si compenetrano (...). Questa visione della natura, con la vittoria della teoria evoluzionistica si è persa. questa è la diagnosi che per noi ne deriva e che oggi appare per lo più inoppugnabile». Ancora, vorrei dire al senatore Pera che l'ultimo autore che si è trovato a commentare nel più recente "Commentario alla Costituzione" l'articolo 2, il professor Emanuele Rossi, che l'ha commentato molto bene, ha scritto proprio nei giorni scorsi su un quotidiano queste parole: «(...) quando un ordinamento ha fatto proprio il principio della separazione dei poteri, le "scelte tragiche" sono affidate alla responsabilità di tutti questi poteri, ciascuno nel proprio ruolo, ed è proprio il rispetto del ruolo istituzionale da parte di ciascuno che consente di individuare le scelte che in quella circostanza vengono ritenute migliori e che tali possono anche non essere in base alla morale di alcuni o di molti, ovvero al diritto "naturale" o ad altri criteri con cui ciascuno può legittimamente aderire, ma che nondimeno sono quelle "giuste" per l'ordinamento che le ha adottate. In altri termini, a nessuno è consentito di sostituirsi agli altri poteri anche nell'ipotesi in cui ritenga di essere nel giusto e che gli altri stiano sbagliando». Evitiamo quindi di delegittimare la Costituzione con richiami esterni. Certo, è facile eccitare gli animi, è facile intervenire per esporre teorie che eccitano le platee e soprattutto quelle della propria parte; speriamo che questo non accada più. Ma noi, che manifesteremo per la Costituzione non per annetterci la figura del Presidente della Repubblica o per imbalsamarla, vogliamo appunto richiamare questo spirito. Vorrei terminare con un'ultima citazione, quella del più grande statista del secolo scorso, Alcide De Gasperi, che ci richiama a questo dovere che ogni Presidente del Consiglio dovrebbe imitare. Alcide De Gasperi, andandosi a presentare alla Settimana sociale dei cattolici del 1945, disse: «Avvicinarsi a questa assise è come eseguire una grande ascensione montana: ci si trova in una atmosfera ossigenata. Non sempre, quando si scende dall'alta montagna, è possibile mantenere la stessa atmosfera e direi non sempre la stessa prospettiva può essere attuata, quando si tratti di dover fissare una pratica di convivenza civile

dopo aver sentito l'intervento di un uomo che stimo molto, il senatore Ceccanti, mi sono preoccupato perché la sensazione è stata che abbia sbagliato provvedimento o Aula.

forse stamattina pensava di andare all'università per svolgere la sua lezione e invece è capitato al Senato. Probabilmente nella sua agenda si è creata confusione. Caro senatore Ceccanti, l'abbiamo ascoltata comunque volentieri. Però, lei ricorderà il "*si parva licet componere magnis*"; qui siamo nel *parva* e non nel *magnis.* C'è poi - lei lo ricorderà - una stupenda poesia di Marziale che critica un avvocato il quale, dovendo disputare intorno alla proprietà di tre caprette, parla citando Giove, Minerva, Marte e così via, e alla fine il poeta dice: "Bene, tonitruante patrono, vieni adesso alle tre caprette".

Fuori di questa schermaglia che ritengo amabile e che dovrebbe improntare il più spesso possibile i lavori parlamentari, mi pare addirittura di poter dire che vi era in me l'aspettativa di un voto favorevole dell'opposizione a questo provvedimento. Questo lo dico per il lavoro intensissimo fatto in Commissione (e ringrazio il presidente Vizzini e il relatore Malan), per la costruttività

Invece, l'ansia di contrapposizione comunque vi ha fatto valutare non l'insieme di questo provvedimento, ma alcuni punti che non vi piacciono e che enfatizzate diventando ciò la scaturigine per far sì che la vostra sia una posizione di contrasto e di voto contrario. Speriamo che le cose cambino e che quando si arriva ad un milleproroghe, dove vengono accolti tanti emendamenti dell'opposizione, dell'opposizione, l'opposizione capisca che quando noi siamo all'opposizione facciamo i ragionamenti che fanno loro oggi e, viceversa, se loro torneranno al Governo riprenderanno questi stessi ragionamenti, che sono sempre gli stessi: la necessità, l'urgenza, l'articolo 77, la decretazione, la congruità rispetto alla possibilità per la Corte costituzionale di entrare nella valutazione dei requisiti, l'enorme numero di decreti, la fiducia; tutte cose che io per due anni alla Camera ho ripetuto tutti i giorni e che adesso sento ripetere qua, sono sempre le stesse. Il ministro Vito è un grande esperto di procedura parlamentare e sa che quanto sto dicendo è esattamente la verità. Dunque, sgombrato il campo da tutto questo e rimanendomi poco tempo a disposizione, le ragioni per le quali si è posta la fiducia sono quelle che ho appuntato quando ha parlato il ministro Vito: i tantissimi emendamenti (oltre 400), i tempi brevi, i sessanta giorni della decretazione d'urgenza e, soprattutto, il rispetto per il lavoro in Commissione, perché non dobbiamo dimenticare che quasi tutti gli emendamenti parlamentari sono stati inseriti nel maxiemendamento maxiemendamento governativo. Il che vuol dire rispetto per un Parlamento che ha lavorato tanto, seppur in Commissione, e non negazione del dibattito, né in Commissione, né in Aula, perché anche in Aula abbiamo ascoltato, sia in discussione generale che nella discussione che nella discussione sulla fiducia, una serie di interventi che hanno ben delineato le posizioni dell'opposizione. Non si dica che non teniamo in pugno la nostra maggioranza e ricorriamo alla fiducia per questo, perché questa affermazione è fuori dal mondo. Se avessimo voluto tenere in pugno la nostra maggioranza avremmo impedito ai nostri senatori di presentare emendamenti. Invece sono più gli emendamenti della maggioranza che quelli dell'opposizione, per quanto abbiamo visto sia in Commissioneche in Aula*. Questo lo dico per paradosso, senatore Morando. È ovvio, non è che non si possano fare delle affermazioni per paradosso; noi certamente abbiamo dei senatori che si sono impegnati e che hanno visto approvati tanti emendamenti. allora sugli elementi positivi di questo provvedimento, non riprendendo argomenti che anch'io ho già affrontato in discussione generale, ma evidenziando i nuovi interventi governativi contenuti nel maxiemendamento. Estremamente importante, lo ricordava il senatore Garavaglia, l'emendamento sugli enti locali, che non sanziona il mancato rispetto del patto di stabilità interno per interventi infrastrutturali ove approvati dal Ministero dell'economia e dalla Conferenza Conferenza unificata, così come i criteri sul pubblico impiego che sono stati introdotti e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa

un'importante norma in materia di detenuti, con cui si permette al garante dei detenuti, che è presente in enti locali o Regioni, di poter accedere al colloquio con i detenuti senza autorizzazione. È questa una norma nuova, che si sposa con quella della quale ho così a lungo parlato ieri e che incrementa, a tutti i costi, la costruzione di strutture carcerarie e paracarcerarie. Infatti, il problema della sicurezza in questo Paese si risolve principalmente costruendo nuove carceri e migliorando il regime di permanenza dei detenuti negli istituti di prevenzione e pena che, come

anche con i soldi della Cassa delle ammende, collega Li Gotti, non sapremo più come difenderci dalla delinquenza. Non possiamo criticare i giudici che applicano la legge Gozzini e che non impongono l'obbligatorietà sostanziale delle misure cautelari quando non sappiamo più dove mettere le persone in stato di detenzione, provvisoria o definitiva, procurando loro disagi da Paese del terzo o del quarto mondo. mondo. Oltre a questo importante emendamento sui colloqui dei garanti dei detenuti, ricordo quali novità la disciplina dei servizi noleggio con conducente; la proroga del termine di applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni; la profilassi internazionale, con i relativi controlli; le importantissime norme sull'editoria; l'Expo di il Fondo unico giustizia, che non è da giudicare in termini di una rimodulazione così negativa come hanno fatto i colleghi dell'opposizione e, da ultimo, la cartolarizzazione degli immobili pubblici, che va a risolvere un problema di grande spessore, in termini, a mio ed a nostro parere, del tutto utili e del tutto congrui. Alla fine di quest'intervento, per tutto quanto ho detto, posso concludere che il Popolo della Libertà voterà a favore della fiducia

è a seguito della fase emendativa e dell'ultimo emendamento del Governo, è molto utile e di buona fattura.

De Luca, De Sena,

Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni,

Franco Paolo Galioto,

Marino Ignazio,

Piscitelli, Pistorio, Pittoni,

sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia: